la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta.

noi pensiamo che sia una misura divisiva che mantiene la precarietà ed, anzi, l'aumenta; non risolve i problemi delle persone e non affronta il problema della povertà.

quelli che prenderanno qualcosa, quelli che prenderanno qualcosina e quelli che non prenderanno nulla, nel senso che avendoli divisi in categorie, i singoli sostanzialmente non prenderanno nulla. Questo a noi appare un tratto sbagliato perché il meccanismo che c'era prima ed è in vigore ancora oggi, il reddito di cittadinanza, certamente presenta delle distorsioni,

credo - non ho alcuna intenzione di giustificare chi sceglie di vivere senza lavorare. Io penso che il lavoro sia un dato importante, però come si fa

Quanto pensate che possano tirar su persone che magari non hanno una professionalità, oppure chi ha la professionalità, perché ha studiato, prende un lavoro così com'è? L'impressione che ho è che voi volete la giustificazione per dire che sono dei poltroni: questo è il dato vero. Una giustificazione per dire

(sindacati e Confindustria), fare insieme una grande discussione su una prospettiva di lavoro e sulle condizioni, invece niente di tutto questo. Avete deciso di comunicare e basta; questo non è un modo di coinvolgere. Comunicare è un fare dispotico: io decido e tu obbedisci.

onestamente, quando ho messo su famiglia, io e la mia compagna lavoravamo in una fabbrica, avevamo uno stipendio e su questo abbiamo costruito il nostro futuro. Mia figlia che è precaria, come fa a costruire questo futuro? Questo è il punto e voi avete introdotto ulteriore precarietà; oltre al salario povero, avete allargato le maglie dei

è proprio questo: una visione, andare in questo indirizzo. Voi non affrontate il problema della precarietà, non affrontate il problema del salario povero e nello stesso tempo non affrontate - visto che parliamo di decreto lavoro - il problema del recupero della perdita del potere d'acquisto. Ora, per fortuna, devo dire che c'è qualche segnale che va in controtendenza - mi avvio alle conclusioni

una senatrice deliziosa, i piccoli rifiuti, ma lei stava peggio di me: i brutti e i belli sono a volte accomunati dall'insolito destino del pregiudizio.

"persino io", non lo dico per me e non c'è rabbia per una lesa maestà. Sono un po' contro le maestà e non me ne voglia qualcuno, ma verifico e condivido con voi - che in questo periodo siete parte della mia famiglia di ideali, anche se talvolta come sia ancora grave la situazione del pregiudizio legato alle disabilità. Certe volte persino una pacca sulla spalla può risultare offensiva piuttosto che di aiuto.

positività per il provvedimento e, in alcuni punti, anche la mia soddisfazione, soprattutto per ciò che riguarda le disabilità. Mi sembra che anche molti senatori della minoranza abbiano colto la sfida positiva del provvedimento, sia in Commissione, sia in

che solo qualcuno ha ragione e gli altri hanno tutti torto, cosa che spesso sento dire, ohimè, anche in quest'Aula: da psichiatra dico che, o è una cattiva politica, o addirittura è una malattia mentale, perché chi pensa di avere sempre ragione solo perché è schierato dall'altra parte "toppa forte" oppure è in contraddizione con il proprio

sentirmi sempre dalla parte della ragione. La ragione c'è quando viene condivisa, anche in parte,

la vera conquista bella è quando si condivide con l'avversario una sfida. Per me questo provvedimento è proprio sotto questa

il lavoro è parte integrante, fondamentale, irrinunciabile completamente costitutiva del nostro io. Si può vivere senza amore, anche se mi auguro che nessuno di noi viva questo. Ringraziando entità superiori e non la mia capacità, sono sempre stato amato, anche stamattina e fa bene alla salute, ma il lavoro è precondizione di ogni cosa, sia quando si vive, che quando si lascia per anzianità. Purtroppo - e lo dico anche per il lavoro è molto spesso un sogno che parte da lontano e arriva forse troppo tardi; qualche volta per qualcuno

Luciano Violante, un tosto, ma onesto Presidente della Camera, celebrando il 1° maggio come quest'anno: per molte categorie di persone, che rappresentano il Sud del Sud, le persone con disabilità, il lavoro è spesso tramutato in un incubo per la lunghezza, per il dileggio, per la disconferma di chi ti dovrebbe dare lavoro

superare in parte tale incubo. Dico in parte, perché non si possono fare le nozze con i fichi secchi (e qui non ci sono né nozze, né fichi secchi). c'è la volontà del Governo e di una parte più ampia della maggioranza (per fortuna), anche fuori dal Senato e dalla Camera, che vede questa sfida lavoro come una sfida colta positivamente, anche se certo con difficoltà. È un periodo complicatissimo; chi non lo riconosce o non vede quello che compare o è un cretino. Essendo psichiatra, me lo posso permettere, perché me ne intendo, magari del cretinismo mio, che vi giuro non è voluto, ma è naturale; ognuno decade un po' ogni anno nella propria cerebralità. Mi avvio alle conclusioni. Credo che le critiche servano più delle vitamine, sicuramente più dei vaccini, dei quali spesso stra-abusiamo. Però le critiche devono essere coerenti, perché non noi nel Senato, ma i cittadini hanno più bisogno di verità che di qualsiasi altra cosa. Le bugie fanno male alla salute della democrazia. Io credo che le critiche serie siano dolorose, perché quando si critica

certo criticando anche tra di noi, magari non con la mancanza di puntualità (ma lasciamo stare). Credo che un provvedimento - concludo, Presidente, e mi scuso

con chi non la pensa come noi, perché la democrazia, perché la legge, perché l'emendamento, perché la pacca sulla spalla vivono se noi le condividiamo, altrimenti è solo una lotta sterile, che non ha senso

al lavoro degli altri, anche se sinceramente lavoro ancora, perché lo considero un miracolo per me, perfino un dono meraviglioso. Continuo a farlo con il massimo della gioia, anche quando magari sbaglio, quando mi dicono che sbaglio o che scoccio, come adesso. Lo considero sempre una meraviglia, soprattutto il lavoro vero, quello scelto, e possibilmente condiviso con le persone che la pensano come noi o al contrario di noi, ma condividono questa sfida.

il mercato del lavoro italiano non gode di buona salute, sono ormai enormi le sacche di precarietà, per cui dopo cinque anni solo pochi giovani riescono a passare a un contratto stabile. Il fenomeno delle false partita IVA presenta numeri sempre più in crescita e troppi sono i contratti atipici. C'è poi il problema dei bassi salari: rispetto alle retribuzioni medie dei Paesi OCSE, l'Italia si piazza al ventitreesimo posto su 34 Paesi, con salari reali che dal 2012 sono rimasti immutati, allo stesso livello, mentre in Francia e in Germania sono cresciuti di quasi il 20 A sottolineare la drammaticità di questo fenomeno, richiamo il dato secondo il quale circa 3 milioni di lavoratori, pari al 15 per cento della forza lavoro complessiva, hanno retribuzioni tali da vivere sotto la soglia di povertà e non finisce qui, purtroppo. L'intelligenza artificiale e la crescente automazione dei processi produttivi presto scuoteranno dalla base il mondo del lavoro per come l'abbiamo conosciuto fino adesso; interi settori cadranno in disuso e altri ne nasceranno e la maggior parte dei lavoratori sarà chiamata ad acquisire competenze per svolgere mansioni profondamente diverse da quelle che adesso svolgono. Dall'altro lato, si impone il carovita: nel 2022 il costo della vita è cresciuto di sette punti e le retribuzioni invece appena del 4 per cento, gli affitti sono esplosi e non parliamo degli interessi sui mutui. E allora, davanti a uno scenario del genere, questa attesa riforma che prende il nome di «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro», tanto preannunciata come la fine dell'assistenzialismo generato dal reddito di cittadinanza, non mi sembra che colga nel segno delle reali necessità dei lavoratori, lasciando scoperte le caselle più importanti: il salario minimo, la stabilizzazione del rapporto di lavoro, la sicurezza dei luoghi di lavoro, la formazione professionale e, in ultimo, il cuneo fiscale. Sulle Sulle retribuzioni si continua a fingere che tutto vada bene, ma anche Confindustria ha detto chiaramente che bisogna introdurre il salario minimo per contrastare il fenomeno del lavoro povero c'è nulla che favorisca la stabilizzazione dei contratti, ma ancora una volta si vara una norma a vantaggio dei contratti atipici e dell'espansione del ricorso ai *voucher*, visti quale strumento per allargare le maglie del lavoro stagionale a discapito di una politica di lavoro che invece dovrebbe investire sui settori produttivi più interessati dalla stagionalità, favorendo la flessibilità del lavoro ma senza rinunciare alla stabilità dell'occupazione. In questo senso, aumentare la possibilità di ricorrere ai *voucher* non significa creare lavoro, ma legittimare i datori di lavoro a ricorrere all'impiego di forza lavoro senza alcuna tutela. E che dire poi delle politiche per favorire l'occupazione femminile, grandi assenti di questo provvedimento che ha visto presentare solo proposte in Commissione per alleggerire le sanzioni a carico delle imprese che non versano i contributi ai lavoratori? interviene anche contro le morti bianche, una vera emergenza del nostro Paese. Lo scorso 6 giugno l'INAIL ha pubblicato i dati relativi agli infortuni sul lavoro del primo quadrimestre 2023;

A fronte di una situazione così drammatica, non si registra un impegno concreto per contrastare questo fenomeno e anche ieri sera il Governo ha nuovamente espresso parere contrario all'emendamento con il quale si chiedeva di mettere a disposizione le risorse per i dispositivi di autospegnimento e segnalazione delle anomalie dei macchinari

Il provvedimento invece interviene in maniera importante sul reddito di cittadinanza, decretando la sua fine e la sua sostituzione con due strumenti che prenderanno il nome di reddito da inclusione e reddito da lavoro. È vero che il reddito di cittadinanza andava migliorato, in particolare nella parte relativa alle politiche attive per contrastare gli abusi che hanno finito per creare un effetto distorsivo sul mercato del lavoro, ma proprio per tale ragione era questa l'occasione per introdurre finalmente il salario minimo

stessa - in cui si stabilisce che ogni lavoratore ha diritto a una retribuzione che non solo deve essere proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, ma che deve anche garantirgli un'esistenza libera e dignitosa. Invece, avete introdotto un meccanismo a collo di imbuto che avrà come unica conseguenza la perdita del sussidio per numerose famiglie. Avete previsto l'obbligo per il lavoratore di accettare l'offerta di lavoro, pena la perdita del reddito da lavoro, senza limitazioni di distanza tra la sede in cui quel lavoratore vive ed ed il luogo in cui dovrebbe andare a lavorare, introducendo una disposizione che ha una natura ricattatoria, perché prevede che, al rifiuto, questi perderà anche il reddito. Una disposizione lesiva, indubbiamente lesiva, della dignità del lavoratore e dell'individuo. L'idea che una famiglia, per accettare una qualsiasi offerta di lavoro, si debba trasferire anche a mille chilometri da casa è un'idea che sta fuori dalla realtà, soprattutto quando, a fianco di questa disposizione, non avete accettato di fissare la soglia minima della retribuzione oraria. Con i nostri emendamenti, respinti sia in Commissione che in Aula, dove li abbiamo riproposti con tenacia e con convinzione, avevamo previsto di fissare tale soglia di retribuzione oraria a 9 euro lordi. Io mi domando come pensate sia possibile che un lavoratore si trasferisca in un'altra città senza prevedere che aumenteranno i costi necessari per vivere, per procurarsi un alloggio, per trasferire la sua famiglia, per il trasporto, per le prestazioni essenziali come l'istruzione e la sanità. Signor Presidente, in Commissione tutte le forze di opposizione hanno lavorato in modo coordinato e congiunto per tentare di migliorare questo provvedimento. La gran parte delle proposte che abbiamo presentato, però, sono state respinte, come quella per aumentare la dotazione del fondo per l'assegno alle vittime di violenza e quella per aumentare la dotazione per la tutela delle famiglie con disabili e per tutti quegli altri contesti di estrema fragilità che avevano trovato, nel reddito, un elemento di sostegno. Su tutte queste misure, ci è stato risposto che non c'era copertura finanziaria. Signor Presidente, altri Paesi europei, invece, si stanno attrezzando per prepararsi all'enorme trasformazione del mercato del lavoro con riforme ben più sostanziose. La Spagna, ad esempio, ha approvato una riforma che rende i contratti a termine l'eccezione, principio già sancito, peraltro, dalla Corte di giustizia europea, che ha condannato l'Italia per il ricorso immotivato al lavoro a tempo determinato anche nella pubblica amministrazione. La Germania ha approntato un piano di riforma del reddito di cittadinanza, per cui i beneficiari non saranno più indirizzati verso il primo lavoro disponibile, ma collaboreranno con i centri per l'impiego in un percorso di formazione per il lavoro a tempo indeterminato. Anche l'Italia dovrebbe imboccare questa strada: lavoro pagato il giusto, riduzione dei contratti atipici, formazione permanente per occupati e disoccupati. È l'unico modo per reggere l'urto delle grandi trasformazioni tecnologiche, che avanzano, che arrivano. Non possiamo voltarci dall'altra parte, pensando che questa riforma le fermerà o comunque le mitigherà. Quello, quindi, che ci preoccupa di più è la constatazione che il Governo continua a avere un approccio vecchio, assecondando quel falso mito secondo il quale il mercato del lavoro funziona male perché è troppo rigido. In verità, sono vent'anni che il mercato del lavoro è stato reso flessibile in ogni modo, aprendo il ricorso generalizzato a contratti a tempo determinato e introducendo quelle figure atipiche di lavoro parasubordinato che hanno dato origine alle false partite Iva e creato una generazione di precari del lavoro e della vita. In conclusione, signor Presidente, non ci riteniamo soddisfatti da questo provvedimento, che non ha affrontato i temi cruciali del lavoro e ha introdotto nuove disposizioni che non risolveranno la crisi occupazionale, ma aggraveranno la situazione di tantissime famiglie, generando solo nuove povertà. Per onestà intellettuale, riconosciamo al Governo il merito per l'intervento sul costo del lavoro, anche se risulta evidente che il taglio provvisorio del cuneo fiscale è insufficiente rispetto all'aumento del costo della vita. Però, cogliamo il segno di un indirizzo politico corretto e su questo esprimiamo sinceramente la nostra condivisione. Così come condividiamo ed apprezziamo la proroga del lavoro agile per i dipendenti fragili della pubblica amministrazione, ringraziando la senatrice Mancini per avere fatto propria la misura e proponendo il relativo emendamento. Prendiamo infine atto, e di questo ringraziamo maggioranza e Governo, dell'approvazione degli emendamenti a tutela delle competenze delle autonomie speciali nelle materie al centro del provvedimento, ribadendo la necessità della tutela delle autonomie, che costituiscono espressione del loro territorio. In virtù di questi elementi, ci sembra evidente che le luci di questo provvedimento non riescono comunque a superare le numerose ombre che le nuove disposizioni getteranno sul mondo del lavoro. Per questo, annuncio il voto di astensione del Gruppo Per le Autonomie.

colleghe e colleghi, prima di tutto desidero ringraziare i Presidenti delle Commissioni 10a e 5a, il presidente Zaffini e il presidente Calandrini,

Sul primo punto il nostro giudizio è chiaramente positivo, però osserviamo alcuni punti di criticità. In particolare permangono forti dubbi sull'effettivo funzionamento delle politiche attive, che fino a oggi, anche da prima del reddito di cittadinanza, non hanno funzionato affatto e su questo chiederò e chiedo un'attenzione particolare del Governo. Come ha scritto qualche giorno fa il professor Seghezzi, tutto ad un tratto si affida completamente la sopravvivenza di centinaia di migliaia di persone al fatto che troveranno un corso di formazione che non solo lo troveranno, ma lo troveranno subito. Inoltre, se già è difficile dare per scontato che si verrà inseriti rapidamente in uno dei corsi appena indicati, ancora più difficile è immaginare che questi portino automaticamente a trovare un lavoro. È evidente che anche su questo noi chiediamo una maggiore attenzione, perché sul presente decreto-legge bisognava fare un investimento maggiore. Il secondo punto concerne il cuneo fiscale.

come abbiamo evidenziato anche con i nostri emendamenti. Certamente ci sono misure che noi consideriamo altrettanto positive, quali, ad esempio, l'estensione dell'assicurazione INAIL agli studenti, l'obbligo di nominare il medico competente ogni qualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza; l'estensione ai lavoratori autonomi delle misure di tutela per la salute e la sicurezza previste nei cantieri temporanei; l'incremento di alcune misure di sicurezza sul lavoro.

pensando a Luana D'Orazio, a quella ragazza che due anni fa ha perso la vita proprio in un luogo di lavoro. *(Applausi)*. Chiedevamo di mettere finalmente a sistema una normativa di civiltà,

economicamente, di non avere paura di denunciare il proprio compagno violento. Quindi si tratta di un grande emendamento per il quale ringraziamo certamente il Governo e tutte le colleghe e i colleghi che lo hanno sottoscritto. Ma si doveva fare di più, poiché c'era anche un'altra proposta emendativa, volta ad aumentare le risorse del Fondo per il reddito di libertà di 40 milioni di euro in due anni. Queste sono delle priorità. Il pasticcio di ieri in Commissione bilancio evidenzia che questa maggioranza è andata completamente in *tilt* e noi non potevamo certo essere la stampella di questa maggioranza ma abbiamo evitato il peggio perché consideriamo alcuni provvedimenti contenuti in questo decreto-legge importanti, anche perché frutto di un lavoro che abbiamo fatto anche con il Governo Draghi, insieme a colleghe e colleghi nella scorsa legislatura.

particolare le colleghe e i colleghi del PD e dei 5 Stelle che hanno sottoscritto anche molti dei nostri emendamenti - per evitare il peggio ieri in Commissione bilancio, evitando appunto che si lasciassero risorse su provvedimenti sicuramente non prioritari *(Applausi)* rispetto alla sicurezza nei luoghi di lavoro, rispetto alla violenza di genere e al reddito di libertà. Per tutte queste ragioni noi pensiamo che si poteva fare di più, perché i criteri dovevano essere quelli della universalità, dell'equità e dell'efficienza, doveva essere il provvedimento delle misure strutturali. Penso anche al tema dei lavoratori fragili, dei lavoratori con disabilità. *(Applausi)*. Ieri la collega Versace

Saremo sempre al vostro fianco fino a quando questi importanti temi che riguardano la sicurezza nel mondo del lavoro saranno portati finalmente in un sistema strutturale di misure che non dovranno essere più ricercate nelle leggi di bilancio.

Su opzione donna avremmo voluto sentire delle parole molto più chiare. Anche dalle audizioni sono emerse richieste esplicite da parte di tutte le categorie; allora perché non ascoltarle? È evidente che non si può

delle due carte. Per tutte queste ragioni, evidenziando i lati positivi e negativi di questo provvedimento, noi che siamo un'opposizione costruttiva, propositiva e che fino all'ultimo ieri abbiamo cercato di lavorare con proposte emendative chiare, ci asterremo come terzo polo, come Italia Viva e Azione, augurandoci però che la maggioranza possa trovare risorse aggiuntive su un tema così importante come quello del lavoro.

con un impianto che è sostanzialmente confermato dal lungo esame parlamentare; in questo caso mi rivolgo alla Commissione lavoro del Senato e alla relatrice, che ringrazio per il lavoro svolto. Sempre in Commissione è continuato e proseguito il vastissimo ascolto delle parti sociali. Non si dica quindi che questo decreto-legge nasce in solitudine e in autonomia, dalle menti di qualcuno.

Viene aumentato di 4 miliardi il taglio al cuneo fiscale, che porta il totale a 7 miliardi, posto che già la legge di bilancio di dicembre aveva iniziato giustamente questa strada. Ora il taglio per i redditi fino a 25.000 euro vale complessivamente 7 punti percentuali e un lavoratore può avere un beneficio in busta paga fino a 100 euro mensili; non credo sia poco. Per i redditi fino a 35.000 euro il vantaggio fiscale è complessivamente pari a 6 punti percentuali. In questo modo il Governo e la maggioranza dimostrano una particolare attenzione ai redditi medio bassi, mettendo in campo risorse adeguate; anche questo non è mai stato scontato. La conferma del taglio del cuneo, che pesa circa il 45 per cento sul costo del lavoro, è tra l'altro uno degli impegni elettorali del centrodestra. La sfida ora è quella di rendere strutturale questa misura trovando le risorse finanziarie entro la prossima legge di bilancio. le risorse possano venire sia dalla crescita dell'economia che da una puntuale lotta all'evasione fiscale. L'attenzione alla necessità dei lavoratori con redditi medio bassi viene però anche confermata dalla possibilità di utilizzare i *fringe benefit* aziendali per il pagamento anche delle utenze domestiche. L'idea di ridurre le tasse sul lavoro prosegue attraverso una serie di altre disposizioni del decreto-legge; una misura che detassa il lavoro notturno e festivo per i dipendenti delle strutture turistico-alberghiere, una maggiore flessibilità per le prestazioni occasionali nel settore turistico e termale; viene incentivata l'inclusione di lavoratori con disabilità che abbiano meno di trentacinque anni; vengono semplificate le informazioni e gli obblighi per il datore di lavoro, togliendogli quindi quegli oneri che rappresentano sempre un costo; anche questo è un aspetto poi un'attenzione particolare all'inserimento e al reinserimento nel mondo del lavoro; vengono appostati un miliardo e 350 milioni per la formazione, introdotti incentivi pari al 60 per cento della retribuzione lorda per l'assunzione di giovani sotto i trenta anni di età, di età, reso più fruibile il contratto di lavoro a termine, che ora potrà essere rinnovato fino a ventiquattro mesi in presenza di ragioni tecniche, produttive e organizzative. alle aziende interessate dai contratti di espansione di gruppo per completare il *turnover* previsto, viene consentito ai lavoratori più anziani di uscire in un arco temporale più ampio; la misura è importante perché all'uscita dei lavoratori anziani dovrà corrispondere l'assunzione di nuovi lavoratori. Questa è una richiesta che viene anche dal mondo produttivo. Viene consentito agli enti del terzo settore di attingere a specifiche competenze in deroga al limite retributivo previsto. queste le principali misure previste in tema di lavoro che si uniscono ad altre disposizioni puntuali ed anche settoriali, a salvaguardia di posizioni lavorative o contributive. C'è poi l'ampio capitolo, affrontato da tanti colleghi, delle disposizioni che riguardano l'istituzione dell'assegno di inclusione. È importante, perché dopo quattro anni in cui si è fatto credere che potesse esistere un reddito, non da lavoro, ma di cittadinanza, si cambia registro, com'è giusto che sia. Si introduce una misura per contrastare la povertà, sì, e al contempo si delinea il campo dei soggetti che possono accedervi. Il reddito di cittadinanza, tra l'altro senza limiti di tempo, non è riuscito a coniugare i due scopi per cui era stato concepito: contrasto alla povertà e politiche attive. Lasciava fuori troppi poveri veri e veniva elargito in troppi casi ai cosiddetti furbetti. I meccanismi del passaggio tra la percezione del beneficio economico e l'inserimento nel mondo del lavoro erano tortuosi e gestiti da strutture pubbliche e purtroppo inadatte allo scopo. Questo, purtroppo, è stato dimostrato. Non solo non ha funzionato la parte delle politiche attive, ma è stato spesso un disincentivo al lavoro: questo nel nostro Paese non possiamo permettercelo. La nuova misura ha parametri differenti e un sistema di controlli più articolato. Sono previsti filtri ulteriori sia al momento della richiesta dell'assegno, sia al mantenimento dello stesso, che prevedono la verifica sulle banche dati dei requisiti richiesti. Al contrasto della povertà e all'inclusione vengono destinati 5,5 miliardi, a partire dal 2024, mentre il reddito di cittadinanza finisce a dicembre di quest'anno. Ma era necessario, colleghi, ridisegnare fin d'ora la nuova misura e dotarla di una copertura adeguata, posto che l'assegno di inclusione avrà il doppio della dotazione del reddito di inclusione, quella misura che aveva preceduto il reddito di cittadinanza. Quindi, l'assegno di inclusione adesso andrà solo a coloro che ne hanno veramente bisogno e contiamo che questo possa davvero accadere fino in fondo. Per inserire o reinserire nel mondo del lavoro chi non lo ha, vengono ridisegnati anche i percorsi delle politiche attive, per il supporto e la formazione alle persone tra i diciotto e i cinquantanove anni. È un decreto, insomma, molto articolato che affronta molti punti in tema di lavoro e protezione sociale, con l'intenzione di risolvere quelle criticità che sono emerse dall'applicazione della normativa vigente. Certo, colleghi, non si risolvono tutti i problemi del mondo del lavoro e della povertà. Però, lasciatemelo dire, soprattutto viene ridato al lavoro quel tono di dignità che il lavoro merita, meritava e che dobbiamo continuare a tutelare. I senatori del Gruppo di Forza Italia hanno partecipato ai lavori della Commissione lavoro e hanno visto accolte anche alcune delle proprie proposte per migliorare il testo. Anche per questa ragione, quindi, è con convinzione che dichiaro il voto favorevole del nostro Gruppo.

«misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro»: è questo, almeno a parole, l'obiettivo di un decreto-legge che il Governo ha strumentalmente approvato il 1° maggio, trasformando anche la festa dei lavoratori in un'occasione di divisione e non di unione del Paese. Abbiamo creduto, in modo romantico devo ammetterlo, che con tale provvedimento urgente, l'ennesimo da quando l'Esecutivo è in carica, si sarebbe preso di petto il tema dei salari bassi, ad esempio con il salario minimo: un'assoluta priorità in questo Paese, in cui negli ultimi trent'anni questi sono diminuiti. Ancor di più oggi, con l'aumento dell'inflazione e delle rate dei mutui, che sta mettendo a dura prova le famiglie italiane, veramente c'è bisogno di alzare gli stipendi. Con questo decreto non solo non rispondete alle reali necessità e urgenze dell'Italia, ma anzi si va in direzione opposta, rendendo sempre più precario il mondo del lavoro e penalizzando le categorie più fragili. Tutto per fare un po' di cassa, tutto solo ed esclusivamente per assecondare il consenso elettorale. *(Applausi)*. Veniamo ai contenuti di questo decreto-legge: la sostituzione del reddito di cittadinanza con una nuova misura di inclusione sociale. Ve lo devo dire: alla fine, dopo anni di insulti e attacchi sguaiati, siete riusciti a comprendere l'importanza di questa misura, visto che avete praticamente copiato il suo impianto, traslandolo nel vostro nuovo strumento. Non potevate però non dare sfogo alle falsità che avete propalato in campagna elettorale. Dunque, lo avete peggiorato, al punto da penalizzare le categorie più fragili. Siamo passati da una misura universale di contrasto alla povertà, come il reddito di cittadinanza, ad una che discrimina le famiglie sulla base di criteri che prescindono da quelli economici: i figli, le disabilità, la presenza o no nel nucleo di una persona anziana. Siamo il primo Paese in Europa a fare questo e, almeno su questo, un primato lo avete raggiunto. *(Ilarità).* In Commissione avete dimostrato di avere le idee confuse e per fortuna che dicevate di essere pronti! *(Applausi)*. Il testo uscito dal Consiglio dei Ministri escludeva i senza fissa dimora, le donne vittime di violenza e molti altri soggetti fragili, dalla possibilità di percepire il nuovo assegno di inclusione. Una follia! Con un emendamento avevamo chiesto di inserirli tra i beneficiari. Avete provato a farlo, approvando un vostro emendamento, ma per le coperture finanziarie siete andati a modificare la scala di equivalenza a svantaggio dei disabili. Ieri pomeriggio abbiamo visto tutti quello che è successo. Probabilmente vi siete accorti della malparata e, con un emendamento della relatrice, avete corretto il tiro, non dopo comunque aver presentato anche un emendamento per aumentare le spese della comunicazione di Palazzo Chigi, e questo è scandaloso. Siete ridicoli. Togliete i soldi ai disabili per darli ai fragili, per poi riportarli ai disabili, e darli poi a Palazzo Chigi. Dopo tanto "togli e metti", l'unica cosa intoccabile in questo decreto-legge sono le spese per finanziare l'acquisto di armi. Avete poi fatto retromarcia sul nostro emendamento per la detassazione delle assunzioni delle badanti e, anche in questo caso, avete fatto tutto da soli. Peccato che poi alla fine le famiglie siano rimaste illuse da questa cosa e poi deluse, quando in Commissione bilancio avete tolto tutto. Avete deciso che le famiglie con figli sopra i quattordici anni possono essere separate, perché il padre, ad esempio, sarà obbligato ad accettare un lavoro in Lombardia, mentre il resto della famiglia resterà a vivere in Calabria. Per fortuna che eravate quelli a favore della famiglia! Andiamo avanti con lo *smart working* per i fragili: sì nel settore privato, no nel settore pubblico e ora, in Aula, sì, ma solo fino a settembre. Anche qui è chiaro, che per voi, i dipendenti pubblici rappresentano un peso per lo Stato e non una risorsa da valorizzare, visto che nel DEF non avete messo un euro per il rinnovo il rinnovo dei contratti. Cosa dire delle politiche attive del lavoro, dove il detto "la mano sinistra non sa cosa fa la destra" calza a pennello? Avete ereditato i soldi del PNRR per la formazione, 4,4 miliardi di euro per l'attuazione del programma GOL e per il piano nazionale delle nuove competenze, più 70 milioni di euro per le assunzioni nei centri per l'impiego, un passaggio ineludibile per potenziare queste strutture e renderle più efficienti e moderne. Ebbene, le Regioni, tre quarti delle quali sono amministrate da voi, hanno assunto meno della metà degli 11.600 nuovi operatori previsti. È una follia anche questa. anche questa. Alla fine dello scorso anno, addirittura, Basilicata, Calabria, Molise e Sicilia erano ferme a zero assunzioni. Questo non è possibile. *(Applausi)*. Poi parlate di autonomia differenziata, quando nelle Regioni che amministrate non siete nemmeno in grado di spendere i soldi. colleghi, a noi il disegno è chiaro: state creando un sistema perfetto, che andrà a vantaggio dei privati, a scapito del pubblico e dei fragili. Lo fate con la formazione e con l'inserimento lavorativo, dove le agenzie private avranno sempre più spazio. Lo fate con i servizi pubblici, che puntualmente affidate al privato, facendo proliferare, tra l'altro, l'applicazione dei contratti pirata e del lavoro sottopagato. D'altra parte, è esattamente lo stesso schema che state usando per distruggere la sanità pubblica: dico «state», perché la state distruggendo voi, con i governatori delle Regioni. Le Regioni lo stanno facendo! Tutto questo non potevate non condirlo con quella che voi chiamate flessibilità, e noi invece chiamiamo precarietà e sfruttamento dei lavoratori, con la liberalizzazione spinta dei contratti a termine e dei *voucher*. E chi se ne importa se poi avremo comunque dei pensionati poveri? Fate saltare per legge la causale dei contratti a termine, rimandando la contrattazione collettiva. Ma in che mondo vivete? Vi siete accorti che in questo Paese proliferano i contratti pirata? Ci sono migliaia di persone che lavorano con stipendi bassissimi, di 500 o 600 euro. Ho l'impressione che veramente viviate su un altro pianeta. Lo dico perché, come se non bastasse tutto ciò, in questo decreto, oltre alle causali, autorizzate addirittura la contrattazione *one to one* tra datore di lavoro e lavoratore. Secondo voi, come andrà a finire, quando il lavoratore si troverà davanti un imprenditore che gli propone 500 o 600 euro al mese? Prendere o lasciare. Credo che nessuno di voi abbia mai lavorato un solo giorno in queste condizioni, altrimenti non avreste pensato e scritto tutto ciò.

«Senatrice, le scrivo per farle sapere come siamo stati assunti presso un ospedale pubblico che ha esternalizzato a una cooperativa il servizio di assistenza. Io lavoro presso questo ospedale dall'aprile del 2019; sono stato assunto con un contratto da due ore

Senatrice, come una trentina di colleghi, io prendo 200 euro di tredicesima all'anno, non ci vengono versati i contributi e, quando ci ammaliamo, veniamo pagati per le due ore da contratto. Ci aiuti, senatrice». Questo è ciò che ci chiedono i cittadini. *(Applausi)*. State mettendo alla disperazione migliaia e migliaia di lavoratori. lavoratori. Ve lo dico veramente con il cuore: fermatevi prima che sia troppo tardi. Di fronte a questo grido di dolore non si può restare indifferenti. State facendo le vostre riforme sulla pelle dei lavoratori, rendendo precari nostri giovani: non è giusto. *(Applausi)*. Per concludere, l'altro giorno ho visto molti colleghi della maggioranza commuoversi durante una commemorazione. È legittimo. Concedetemi però un sogno: vorrei vedervi commuovere anche per le migliaia di famiglie che state condannando a una disperata condizione di povertà, per le migliaia di giovani che state condannando alla precarietà Per tutti questi motivi dichiaro il voto contrario del Gruppo MoVimento 5 Stelle.

Finalmente si parla di lavoro e questo il Governo lo fa dal 1° maggio, dalla giornata dedicata al lavoro, e siamo qui per approvare il primo provvedimento dedicato al lavoro.

Non si preoccupi, senatrice, che sui tempi sono molto vigile affinché siano effettivi. proprio per il provvedimento dedicato al lavoro che è stato fatto il 1° maggio. È stato dato un segnale importante, perché abbiamo sicuramente modificato il reddito di cittadinanza. E non ve lo dice una senatrice a caso; ve lo dice la relatrice del provvedimento relativo al reddito di cittadinanza.

soldi che non ritorneranno più nelle casse dello Stato, soldi persi, sprecati, sottratti ai cittadini italiani, come abbiamo ribadito più volte in Commissione e in Aula

Bisognava evitare che la percezione del reddito diventasse un deterrente al lavoro. Molte delle persone che percepivano il reddito cercavano un lavoro, ma volevano lavorare in nero; questo assolutamente andava e va evitato. Lo stillicidio di errori, di mancati controlli e, ancor peggio, di connivenza nel riconoscimento del beneficio o dei buchi... *(Commenti)*. Colleghi, io ovviamente intervengo. Diciamo che, se anche dalla maggioranza si grida, questo non agevola. Lasciate che la Presidenza intervenga, perché al momento è più da questo lato dell'emiciclo che sovrastano le voci. non mi costringete a chiamarvi singolarmente per nome, perché questo ovviamente ha delle conseguenze. Per cortesia, consentiamo alla collega di proseguire senza ulteriori interruzioni. *(Applausi)*. Parliamo allora di statistiche, parliamo di numeri. Solo il 18,8 per cento dei percettori del reddito ha trovato un lavoro, ma non l'ha trovato grazie ai centri per l'impiego; molto spesso l'ha trovato, come succede in Italia, per amicizie o per passaparola. E questo non è politica attiva del lavoro. A decorrere dal 1° gennaio 2024 viene introdotto l'assegno di inclusione, che sostituirà il reddito e la pensione di cittadinanza. Si tratta di un'iniziativa di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, il cui accesso è condizionato alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Oltre ai cambiamenti negli importi e nella modalità di richiesta, ci sono alcune cose importanti che abbiamo introdotto in Commissione.

Abbiamo approvato un emendamento che prevede che i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscano sempre un nucleo familiare a sé, anche per il calcolo dell'ISEE.

fine di evitare gli abusi che ci sono stati fino a adesso. Passiamo quindi dall'assistenzialismo all'assistenza della ricerca del lavoro e all'assunzione stessa. Abbiamo inserito degli incentivi per l'assunzione

ricerca di giovani e di specializzazioni sempre più ricercate, specialmente nell'artigianato e nella meccanica. La continua evoluzione del mercato, la globalizzazione, l'esigenza di far fronte alla stagionalità:

quindi, che anche i rinnovi, e non solo le proroghe di un contratto a termine, saranno senza causali fino a dodici mesi e il contratto può essere, quindi, prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi, e successivamente solo in presenza delle causali. La stessa cosa vale anche per la somministrazione, con l'abolizione dei limiti quantitativi del 20 per cento attualmente previsti per il personale in apprendistato. Questo Governo si occupa anche della sicurezza sul lavoro. Questa mattina abbiamo partecipato alla prima riunione della Commissione d'inchiesta sulla sicurezza sul lavoro e ben venga, ma del tema di occupa anche il Governo direttamente.

contro gli infortuni per studenti e lavoratori della scuola, con la previsione del risarcimento anche per gli infortuni mortali che interessano i giovani in alternanza scuola-lavoro.

privato come una categoria a sé, per poterli reinserire nel mondo del lavoro e fare in modo che abbiano una conciliazione vita-lavoro-famiglia migliore possibile. Infine, parliamo del *welfare* aziendale, uno strumento importante per coprire e garantire servizi che lo Stato non riesce più a garantire e premiare i dipendenti. Le iniziative di *welfare* aziendale agiscono sul livello di *engagement* dei dipendenti, cioè sul loro livello di ingaggio, di motivazione nel lavoro, della loro produttività. Sicuramente serve aggiornare la platea di servizi che possono essere offerti con il *welfare* aziendale sia per la conciliazione vita-lavoro-famiglia della persona, per la genitorialità, ma anche per i *caregiver* o anche solo per l'accudimento dei nostri amici animali. In aggiunta, va aggiornato l'importo dei *fringe benefit*, le famose 500.000 lire poi passate a 258 euro, che poi abbiamo aumentato nel decreto agosto a 600 euro e nella scorsa legge di bilancio a 3.000 euro. Ebbene, ora il nostro Governo ha voluto dare un segnale forte per supportare le famiglie che hanno subìto rincari del costo della vita, del costo dell'energia e del gas, l'aumento dei mutui e la conferma della decontribuzione, grazie al ministro Giorgetti, è un segnale forte della nostra idea di sostegno alle famiglie. Questa è la prima risposta che il nostro Governo vuole dare al mercato del lavoro. Attendiamo il prossimo decreto legislativo sul lavoro. Questo è un primo tassello e sicuramente la risposta della Lega è favorevole a continuare su questa strada, passando dalle parole ai fatti, supportando direttamente i dipendenti sia nel settore privato, sia in quello pubblico, facendo attenzione alla conciliazione sempre più forte del ciclo lavoro-vita-famiglia.

che - a nostro avviso - va immediatamente rilevato. Siete passati, cioè, dall'idea, attraverso *selfie* e progetti mediatici, finalizzata a comunicare questo come un decreto epocale

avete mostrato limiti addirittura nella tenuta della maggioranza. Si sono aperti problemi politici rilevanti all'interno del Governo. Le assenze di ieri non hanno consentito a questa maggioranza di approvare misure sbagliate: avete addirittura provato ad introdurre all'ultimo, senza alcun voto in Commissione, misure inadeguate e improprie rispetto alla compatibilità di questo decreto. Avete cioè provato a portare in Aula un milione di euro da destinare alla comunicazione a Palazzo Chigi, tagliando le risorse per la povertà e favorendo precarietà nel mondo del lavoro.

questa maggioranza. Tuttavia, io voglio segnalare che siete entrati su un piano inclinato. Cominciate a mostrare, anche all'interno della maggioranza, la prevalenza dei ricatti rispetto alle esigenze reali del Paese. che noi intendiamo sottolineare, perché la nostra battaglia non finisce oggi, con il voto contrario a questo provvedimento. La trasferiremo nel Paese, perché siamo sicuri che le dinamiche economiche e sociali che attraverseranno l'Italia e l'Europa renderanno esplicite che le vostre misure, purtroppo, sottendono a un disegno individuale, che non produrrà competitività economica, che lascerà il mondo del lavoro e il mondo dell'impresa dentro tassi di maggiore solitudine e di minore competitività. Questo per noi è il punto cardine della nostra iniziativa politica. *(Applausi)*. Voglio fare due esempi molto semplici, perché noi riteniamo che il sistema di relazioni culturali che attraversa il vostro programma di Governo sia esplicito; abiti altrove rispetto ai valori fondamentali di cui l'Italia e l'Europa avrebbero oggi bisogno per trasformare l'ansia di tantissimi giovani in opportunità e nuova crescita economica. Voglio fare solo due riferimenti: al taglio del cuneo fiscale. Con nostri emendamenti, noi vi abbiamo proposto di impegnare il Governo a renderlo strutturale. Voi avete rinunciato, perché non disponete di alcun progetto per lo sviluppo economico e sociale dell'Italia. Non volete individuare nella lotta all'evasione fiscale un terreno fondamentale per determinare le risorse necessarie per ridurre il costo del lavoro e aumentare i salari. Questa è la questione cruciale. Non potete comunicare o lisciare il pelo all'evasore per ragioni di consenso e poi non individuare le risorse per aumentare i salari e ridurre il costo del lavoro per le imprese che investono in innovazione e in competitività economica, cioè quelle che scommettono sul futuro del lavoro e del nostro Paese. *(Applausi)*. Per noi il lavoro è la questione cruciale, dalla quale dobbiamo partire per fare questo ragionamento. Invece, voi avete una propensione a leggere l'impianto costituzionale del nostro Paese in maniera alternata. Voi avete deciso, in campagna elettorale, di mettere in contrapposizione il reddito di cittadinanza con il tema del lavoro. Come Come dice giustamente l'articolo 1 della Costituzione, il lavoro è certamente un valore fondante della Repubblica, ma vi è anche l'articolo 4, che afferma il dovere di ogni cittadino di svolgere un'attività e una funzione che concorrano al progresso materiale o spirituale della società. Non potete dimenticare però l'articolo 36 della Costituzione, che afferma che il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, in ogni caso sufficiente ad assicurare, a sé e alla famiglia, una esistenza libera e dignitosa.

Voi, invece, con questa operazione nel 2024 porterete l'Italia a essere l'unico e l'ultimo Paese in Europa senza una misura universale per contrastare le povertà *(Applausi)*, perché l'assegno di inclusione che avete introdotto non è un elemento migliorativo del reddito di cittadinanza. Voi avete bisogno delle risorse destinate al reddito di cittadinanza per ridurre il costo del lavoro - questa è la realtà - ma trasformate la povertà in una questione di categorie. Non è così: vuol dire che non avete mai visto un povero *(Applausi)*, perché un povero non necessariamente ha figli disabili e non ha necessariamente più di sessant'anni; un povero, quando vive nel Comune, nel territorio nel quale abita, spesso non ha alcuna condizione di accedere al mondo del lavoro, e dunque anche alla questione della genitorialità, perché ha problematiche che sono spesso di formazione anche psicologiche; ha bisogno di una presa in carico, non di un bancomat, non di un assegno dall'alto. Ha bisogno della presa in carico, che voi negate perché non la rendete più universale e spostate l'attenzione dei servizi sociali, delle comunità, al di fuori delle misure utili per favorire un contrasto concreto alle povertà. La povertà vi disturba: la dovete negare, la dovete lasciare nella solitudine per ragioni di consenso, perché avete aperto una strada sbagliata che mette in contrapposizione la povertà con il lavoro. *(Applausi)*. Cambiate strada e fatelo in fretta! Comunque troverete il Partito Democratico nel Paese a ricostruire la nostra dimensione popolare proprio attraverso tali questioni che non si esauriscono oggi in questo provvedimento sbagliato, lo ribadisco - rischia di spingere l'Italia fuori dalle dinamiche competitive dell'Europa proprio su questo terreno. Chi ci penserà nel 2024 a reintrodurre una misura universale? Noi vogliamo proporlo al Paese, perché con questo impianto culturale l'Italia sbanda e ai giovani e alle famiglie italiane non riuscirete a garantire maggiore sicurezza e maggiore competitività.

dove il tasso di disoccupazione tocca il 22,3 per cento tra i giovani; dove circa il 12 per cento dei lavoratori è in condizioni di povertà; dove ci sono 3 milioni di lavoratori interamente irregolari, serviva serviva offrire misure per trasformare la lotta alla precarietà, indispensabile in questo Paese, come elemento fondamentale per ridurre le disuguaglianze e costruire competitività economica. Voi fate il contrario voi rinunciate ad affrontare il problema dei salari o lo fate semestralmente per ragioni di consenso e ampliate le forme di precarietà, perché sbagliate completamente l'impianto. Lo dico anche alle imprese: non è interesse di un imprenditore che investe sul futuro di questo Paese futuro di questo Paese avere nella precarietà un elemento di competitività; l'impresa ha nella qualità del lavoro l'elemento di competitività per generare futuro e crescita economica. Il vostro modello è sbagliato, siete fuori strada, perché noi abbiamo una gigantesca questione salariale di fronte a noi e una gigantesca bolla di precarietà da contrastare. A me sarebbe piaciuto che questo Governo fosse venuto in quest'Aula anche prima, senza aver bisogno, signor Ministro, di un incidente per il fatto di non avere la maggioranza per i profili finanziari del provvedimento. Questo perché la flessibilità che c'è nel mondo del lavoro ha bisogno di più diritti, non di meno diritti. E avremmo discusso su come aumentare gli elementi di garanzia e di flessibilità. C'è un problema di costo del lavoro e, dunque, c'è un problema di salario congruo alla dignità del lavoro che dobbiamo introdurre in questo Paese, senza il quale cresce la precarietà e non cresce la qualità della buona occupazione. Insomma, avete mostrato di non avere un'idea per il futuro dello sviluppo economico e sociale di questa comunità. Voi privilegiate l'individuo che ce la fa da solo e pensate di costruire crescita lasciando gli altri nella povertà, solitudine e indifferenza di questo Paese. *(Applausi)*. Noi non ve lo consentiremo, perché andremo nel nostro Paese a costruire questa battaglia con i cittadini italiani, per costruire l'alternativa a questa destra.

ovviamente mi fido di lei sull'alleggerimento. Intendiamoci almeno sull'alleggerimento.

10a Commissione ha effettuato. I colleghi erano tutti presenti: ovviamente qualcuno ascoltava meglio e qualcuno ascoltava peggio, ma tutti i soggetti auditi hanno espresso grande soddisfazione per questo provvedimento, ad eccezione - ma lì c'è stato un po' di tasso politico - della CGIL e della UIL, anche se in quel caso abbiamo ascoltato poca materia tecnica e molta materia politica. *(Applausi)*. Comunque ci sono i verbali

presentatori e all'opposizione di discuterli, senza porre la questione di fiducia su un provvedimento che poteva contenere gli elementi

Cito una su tutte che in qualche misura, collega Manca, risponde un po' a tutti i tuoi quesiti. E mi permetto di darti del tu per l'amicizia e la stima reciproca

diciamo che è interessante questa interlocuzione linguistica, e apprezziamo anche l'amicizia,

Colleghi, ne voglio citare anche un'altra. A questo riguardo vorrei anche augurare al collega Magni, che stamattina è stato eletto presidente della Commissione sugli infortuni sul lavoro *(Applausi)*, e alla vicepresidente Testor un proficuo lavoro, Grazie vicenda veramente problematica e fortemente complessa che riguarda la brutta pagina che caratterizza il nostro Paese ormai da tanti anni, ossia l'elevato numero degli infortuni e delle morti sul lavoro, noi abbiamo introdotto nel provvedimento

come dovrebbe lavorare anche il 1° maggio chi è chiamato a rispettare in quel giorno il proprio dovere lavorativo. Per noi quindi è una data simbolica, mentre per voi è divisiva.

Io credo che noi non dobbiamo dimostrare niente. Noi lo dimostriamo dagli atti e dalle azioni di questo Governo. Noi lo materializziamo il nostro non essere omofobi, ma soprattutto ma soprattutto credo che voi non siete in grado di giudicarci. *(Applausi)*. Voi non siete in grado di dire quello che noi dovremmo essere, perché noi semplicemente siamo quello che ci vogliono far essere i nostri elettori, quello che ci hanno chiesto i nostri elettori. I nostri provvedimenti sono quelli che attuano il nostro programma. Abbiamo detto che avremmo corretto il reddito di cittadinanza, distinguendo chi poteva lavorare da chi non può lavorare *(Applausi)*, cioè i fragili, e l'abbiamo fatto. Noi non vogliamo essere come voi e non vogliamo che ci dite come dobbiamo essere per somigliare a voi, perché i nostri elettori ci chiedono

al fare opposizione poi, vi parla uno che in questo caso veramente vi può insegnare, perché noi abbiamo fatto sempre l'opposizione. Noi siamo premi Nobel dell'opposizione, perché per anni abbiamo studiato come fare opposizione. *(Applausi)*. Allora, vi vorrei dire, colleghi, che anche per fare opposizione, ricordando che c'è un verbale che trasmette ai posteri quello che voi raccontate e dite, non si può fare a gara a chi la spara più grossa. Bisogna leggere gli atti, bisogna leggere i provvedimenti *(Applausi)*, dopodiché si possono anche commentare negativamente, ma non può essere la gara a chi la spara più grossa, perché c'è il verbale. Il verbale vi tramanda e nel tramandarvi mette in risalto e a nudo tutti i vostri limiti. Tre Governi, due Ministri del lavoro e ci venite a dire che nel lavoro c'è troppa precarietà. chiudo dicendo che per noi la flessibilità non è sempre precarietà, non è obbligatoriamente precarietà. Anzi, la flessibilità dà modo alle aziende di creare lavoro, pagare lavoro e trattenere lavoro.

che quello che è appena successo durante la dichiarazione del presidente Zaffini - a mio avviso - è molto grave. In particolare, è grave l'offesa che il presidente Zaffini, nonostante la sua carica istituzionale, ha rivolto al Gruppo del MoVimento 5 Stelle dicendo che Di Maio era l'unico intelligente del Gruppo. Credo che questa sia una cosa gravissima e chiedo e chiedo che venga preso un provvedimento contro un'offesa gravissima contro un Gruppo e contro una comunità politica. Presidente Castellone, naturalmente la Presidenza ha cercato di disciplinare. Prendiamo atto della sua richiesta.

intervengo per ricordare che Vladimir Vladimirovič Putin è ricercato dal Tribunale penale internazionale dell'Aja per crimini di guerra, per la deportazione di bambini ucraini in Russia. i crimini di guerra commessi dalla Russia in Ucraina sono molteplici - l'ultimo è la distruzione della diga di Kachovka - ma sappiamo dei massacri di civili, spesso anche in fila per andare a prendere del cibo. La serie di crimini, però, non si limita a quelli compiuti in Ucraina, perché nel frattempo in Russia vengono commessi crimini altrettanto gravi. Voglio ricordare il processo farsa che, in questi giorni, si sta consumando a carico di Aleksei Navalny *(Applausi)*, che è sopravvissuto a un a un avvelenamento nel 2020 e sta scontando una condanna a undici anni e mezzo per frode. È rinchiuso in un carcere di massima sicurezza, nel quale non vengono riconosciuti gli *standard* minimi internazionali.

assistere al processo, perché viene trasmesso in *streaming* ma, nel momento in cui Navalny ha preso la parola, la rete è saltata e quindi nessuno sa sa cosa stia succedendo. So che l'ambasciata russa segue i lavori del Senato e voglio dire al Governo russo che il Parlamento italiano non perderà di vista Aleksei Navalny *(Applausi)*, anche se pensate di chiuderlo e seppellirlo dentro una prigione, e con lui altre persone che hanno perso perso la libertà personale, come Vladimir Kara-Murza, condannato a venticinque anni, o il giornalista del "Wall Street Journal" Evan Gershkovich. Sappia il Governo russo che gli occhi della comunità internazionale sono spalancati, e non solo su quello che avviene in

Vladimir Putin, ricercato dal Tribunale penale internazionale, che l'opinione pubblica mondiale non dimentica, che gli occhi nostri, dei nostri Paesi e dell'opinione pubblica mondiale sono aperti. Non pensino che tutto questo accada fuori dallo sguardo del mondo.

avvenga in un contesto di brusio e con un vociare di questo tipo. Glielo devo dire, perché penso che il rispetto reciproco sia un valore, per cui le chiedo cortesemente, dalla prossima volta, di garantire che il nostro senatore Scalfarotto svolga l'intervento in un clima civile dentro quest'Aula, perché è inaccettabile quanto

mi sembrava che comunque le condizioni ci fossero. In ogni caso, prendo atto del suo appunto e mi sentirò ancor più incoraggiata a redarguire i colleghi, come già faccio moltissimo. Presidente, sono assolutamente d'accordo con il collega Scalfarotto, che voglio anche ringraziare per la sensibilità con la quale ha introdotto l'argomento nella nostra Assemblea di oggi. Navalny non può essere lasciato solo e non possono essere lasciate sole le centinaia di prigionieri politici che si trovano, nell'assoluta indifferenza mondiale, a subire qualsiasi violazione in spregio alle più elementari norme di diritto e di umanità. *(Applausi)*. Credo che il collega Scalfarotto in questo momento

a Navalny e agli altri prigionieri politici le condizioni elementari di un processo equo e di una pubblicità dello Non possono esistere motivi di ordine pubblico che impediscano all'opinione pubblica interna e internazionale di capire che cosa capita di capire che cosa capita all'interno delle mura chiuse di un carcere in cui si svolge un processo come quello di cui parliamo, che ha un impatto fondamentale sui diritti delle persone. Grazie dunque al Gruppo

con un regolamento di conti che ci riporta alla realtà dei Gulag che speravamo dimenticata.

su provvedimenti che hanno visto anche delle contrapposizioni e una dialettica, anche marcata, nell'adozione di un provvedimento, emerga finalmente una condivisione così forte e sostenuta su un valore essenziale e su dei principi di riferimento di costitutiva e fondamentale importanza per la nostra Costituzione, per i trattati dell'Unione europea, per la comunità internazionale nel suo insieme, nelle cose più profonde, più vere e più forti che sentiamo e che vengono espresse in quest'Aula. Sto parlando del riferimento, che deve essere costante, sentito e concreto, ai diritti umani, alla libertà, alla libertà di espressione, al pluralismo politico e allo Stato di diritto. Navalny sta patendo delle ingiustizie, delle violenze, delle repressioni inaudite e, ciò nonostante, la sua figura continua a essere un punto di riferimento per l'intero mondo libero, chiamiamolo per quello che è

Navalny non deve essere soltanto un simbolo, ma deve anche poter continuare nel miglioramento di una condizione carceraria che è molto difficile da poter prevedere; è stato detto che la sua salute è in condizioni drammatiche. alla gente che è intorno a lui, così come alle persone che sono intorno ai prigionieri politici cubani o venezuelani o alla situazione drammatica in Iran, a quello che vediamo di volontà repressiva da parte del regime iraniano addirittura contro i rifugiati politici di campo Ashraf.

Questi aspetti devono e possono essere, nei dovuti modi, sempre rappresentati come elementi di forza della nostra politica estera e dei nostri convincimenti. Grazie per questa opportunità. Condivido con molto convincimento quello che è stato detto e mi auguro, a nome del mio Gruppo, che questo segnale forte al Governo, questo sostegno e questo incoraggiamento vengano dati in ogni modo possibile.

che è strettamente collegata allo Stato di diritto. Mi collego al suo intervento sul fatto che i diritti umani non possono e non debbono avere confini.

*(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'approvazione dell'autonomia differenziata è un provvedimento scellerato, che ho già contestato fortemente in quest'Aula in occasione del mio intervento di fine seduta dello scorso 17 maggio, nel quale parlai dello spezzatino d'Italia. Presi in esame le tre materie che sono l'ossatura e lo scheletro di ogni Paese democratico: scuola, sanità, trasporti e infrastrutture, che esaminerò in tre diversi interventi d'Aula. Quest'oggi rifletterò sullo stato della nostra scuola. L'offerta scolastica e formativa del Paese è un'emergenza su cui la politica tutta insieme, opposizione e maggioranza, è chiamata a riflettere. Occorre fornire risposte rapide e concrete, al fine di arginare la crescente sperequazione. un fenomeno allarmante, rafforzato dai dati forniti dai conti pubblici territoriali. L'investimento pubblico per ogni alunno del Sud, negli ultimi tre anni, è arrivato a toccare i 185 euro, contro i 300 euro medi stanziati per gli studenti centro-settentrionali. Nonostante il PNRR recasse l'obiettivo di sanare la sperequazione tra Nord e Sud, ad oggi il divario permane e si registrano nel Mezzogiorno tassi di dispersione scolastica più elevati. Se a un bambino del Centro-Nord vengono assicurate in media 1.230 ore di formazione, un coetaneo del Sud beneficia di appena 1.000 ore, finendo per frequentare in media quattro ore di scuola in meno a settimana. Come poi riportato dalla Svimez lo scorso 13 maggio, la quota del PNRR prevista per l'estensione del tempo pieno e per la costruzione di nuovi mense nelle Regioni meridionali è scesa dal 55 al 40 un dato allarmante che non tiene conto del fatto che ad oggi meno del 25 per cento degli alunni meridionali della scuola primaria frequenta scuole dotate di mensa, contro il 60 per cento nel Presidente, onorevoli colleghi, da questo Esecutivo ci saremmo aspettati un impegno per ridurre questa sperequazione. Ma l'unica risposta fornita dal Governo Meloni è stata quella di concedere ulteriori forme di diseguaglianza, figlie dell'autonomia differenziata, che di fatto non non farà che incrementare i divari educativi, un'aberrazione legislativa che aumenterà il già abissale divario Nord-Sud, per non parlare per non parlare della differenziazione degli stipendi su base territoriale, con l'introduzione di vere e proprie gabbie salariali. Questo il Paese certamente non se lo può permettere e noi del MoVimento 5 Stelle non lo consentiremo

perché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo.